L'elenco dei senatori in congedo e assenti per incarico ricevuto dal Senato, nonché ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicati nell'allegato B al Resoconto della seduta odierna. Comunico che, in data 21 gennaio 2021, è stato trasmesso dalla Camera dei deputati il seguente disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19» il Presidente del Consiglio dei ministri ha inviato la seguente lettera: «Roma, 26 gennaio 2021 Onorevole Presidente, La informo che in data odierna ho rassegnato al Capo dello Stato le mie dimissioni. Il Presidente della Repubblica si è riservato di decidere e ha invitato il Governo a restare in carica per il disbrigo degli affari correnti. Con viva cordialità, *F.to* Giuseppe Conte». La Conferenza dei Capigruppo ha approvato il calendario dei lavori della settimana corrente, in relazione alle dimissioni del Governo. Con le dimissioni del Governo l'attività dell'Assemblea e delle Commissioni del Senato, in coerenza con i principi generali dell'ordinamento costituzionale, è limitata allo svolgimento di attività legislativa correlata a scadenze costituzionali - principalmente i decreti-legge - o di adempimenti inerenti alle proprie prerogative. Le Commissioni sono autorizzate a convocarsi esclusivamente per esprimere il proprio parere su atti del Governo in scadenza, nonché a proseguire le procedure informative già avviate, incluse le audizioni delle Commissioni riunite 5a e 14a sul Piano nazionale di ripresa e resilienza. Per quanto riguarda i lavori dell'Assemblea, la seduta di domani avrà inizio alle ore 9 con il ricordo del centesimo anniversario della fondazione del Partito Comunista Italiano. I Gruppi potranno intervenire per tre minuti. La seduta proseguirà con l'esame del decreto-legge concernente restrizioni connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, già approvato dalla Camera dei deputati. Per la discussione sono state ripartite tra i Gruppi, in base a specifiche richieste, due ore e venti minuti, escluse le dichiarazioni di voto. Gli emendamenti per l'Assemblea dovranno essere presentati entro le ore 19 di oggi.

Signor Presidente, colleghe e colleghi, la piena tutela del diritto delle donne all'autodeterminazione e alla libera scelta in tema di interruzione volontaria della gravidanza è purtroppo nuovamente sotto attacco in Umbria. L'Umbria si appresta a divenire laboratorio delle destre più conservatrici e retrograde, che vorrebbero evitare a livello locale quanto più possibile l'applicazione della legge n. 194, una legge frutto di tanti anni di battaglie e sacrifici delle donne. Noi donne non usiamo le cosiddette pillole abortive come contraccettive, né lo facciamo per capriccio, tantomeno a cuor leggero, come ahimè sosteneva pochi giorni fa in quest'Aula il *leader* della Lega. Le donne hanno diritto all'autodeterminazione e devono essere aiutate a poter scegliere liberamente, non di certo ostacolate, inserendo con furbizia all'interno di quelle che chiamano politiche a favore della natalità meccanismi volti a dirigere le donne verso una sola direzione, quella da loro voluta. A fine novembre scorso le destre umbre hanno presentato una proposta di legge regionale, attualmente ancora in fase di trattazione, per modificare il testo unico regionale in materia in materia di sanità e servizi sociali. Tale proposta di legge è un insulto alle donne di questo Paese. Si parla Si parla di tutela del concepito e di possibilità che ogni donna ha se adeguatamente informata - sottolineo adeguatamente - di avere una conoscenza diretta della propria fertilità, mediante metodi naturali mediante metodi naturali e inoltre istituisce un assegno prenatale finalizzato a fronteggiare i costi legati alla gravidanza e le spese fondamentali nei primi mesi di vita del bambino, come se un figlio fosse un problema legato al periodo di gravidanza e a pochi mesi dopo, anziché ad anni di sostegno sostegno necessari per crescere i propri figli. Come sta accadendo per molte prestazioni del Servizio sanitario regionale, la Lega in Umbria punta ad esternalizzare i consultori verso strutture private, a fare accordi con assicurazioni private per le donne a casa, punta a coinvolgere solo le associazioni *pro* vita. Leggo che la Regione intende promuovere la formazione di nuclei familiari. Anche qui siamo naturalmente nella visione leghista del nucleo familiare. Cosa significa? La Regione organizzerà matrimoni combinati, matrimoni cosiddetti riparatori oppure obbligherà le coppie non sposate a farlo? E che dire delle famiglie arcobaleno, che ormai sono parte delle nostre comunità? Sì, anche in Umbria. In conclusione, Presidente, in Umbria, come in altre Regioni, la Lega prova a imporre la sua ideologia che va contro le conquiste sociali finora conseguite dalle donne, riportando indietro nel tempo di oltre un secolo la loro condizione esistenziale

Signor Presidente, una notizia che fa rabbrividire e fa calare un velo di tristezza infinita su tutti noi: una bambina di dieci anni è morta a Palermo dopo una presunta sfida estrema di soffocamento, promossa e pubblicizzata attraverso la piattaforma *social* TikTok. La procura ha aperto un fascicolo d'inchiesta, ipotizzando il reato istigazione al suicidio. Si ipotizza che il gesto estremo e incontrollato sia stato ispirato da un video sul *web*, una sfida *social* spinta fino alle estreme conseguenze. Un tentativo stupido, ma purtroppo letale di emulazione dell'insano gesto che sfugge al proprio controllo. La piccola è arrivata in ospedale già in condizioni gravissime per arresto cardiorespiratorio e asfissia prolungata; conseguenze del suo strangolamento volontario con la cintura dell'accappatoio attaccata al termosifone di casa. Questa tragedia, dalle prime indagini, sembrerebbe riconducibile ad uno dei folli giochi *social* che si ritrovano su alcune piattaforme. Non più di qualche mese fa lo stesso sgomento ha destato un episodio dalle dinamiche molto simili. La morte suicida di un bambino a Napoli che sembrerebbe collegata ad una manifestazione estrema di coraggio, sempre su una piattaforma *social*. Da questa tragedia non possiamo che richiamare, da un lato, l'importanza fondamentale dei genitori sulla necessità imprescindibile di seguire e accompagnare sempre i figli nelle loro amicizie e nei loro contatti, anche non lasciandoli soli a navigare nel mondo incontrollato del *web* con tutte le sue insidie e le sue trappole. Dall'altro lato, vi è la necessità di controlli più serrati e continui da parte degli organi preposti e di norme legislative più efficaci non aggirabili, capaci di prevenire episodi drammatici come quelli ricordati. Voglio concludere con un pensiero personale e di tutta l'Assemblea, esprimendo vicinanza alla famiglia e rispetto per il loro dolore. I genitori, pur colpiti dall'immane tragedia che ha sconvolto la loro vita, hanno avuto la forza e il coraggio di compiere un atto di profonda umanità e di amore per il prossimo: donare gli organi della piccola Antonella per salvare altre vite umane. Dallo sconforto della loro tragedia potranno nascere tante speranze di vite nuove. il saluto della scuola che Antonella frequentava: «Ciao, per anni ti abbiamo tenuto per mano, ora ti terremo nei cuori». *(Applausi)*.

ha visto la morte di una bambina di diciotto mesi, la piccola Sharon, per mano del compagno venticinquenne di origine rumena della madre, che era al lavoro. Costui ha detto in un primo tempo che la bambina si era tirata addosso una stufetta. La piccola ha avuto un arresto cardiaco non è riuscita a sopravvivere nonostante la rianimazione. L'autopsia avvenuta all'ospedale di Bergamo, ha rivelato una cosa spaventosa: la bambina era stata malmenata e picchiata in più occasioni

è andato nella stanza dove dormiva l'unica donna e ha cercato di abusare di lei tenendola per il collo, minacciandola, palpeggiandola. Probabilmente nella concitazione, la donna è riuscita a chiamare aiuto, quindi questo non signore è stato arrestato - entrambi erano due senzatetto, lui ospite abituale sia della mensa che del dormitorio - ed è stato trasportato in carcere con l'accusa di violenza sessuale aggravata e di lesioni ai danni della donna. Troppe persone rimangono nel nostro Paese a delinquere laddove non hanno alcun titolo per restare, ma è fortissima la preoccupazione riguardo alla sicurezza

di poter creare una componente in Senato con lo strumento giuridico di base di Alternativa Popolare che ha espresso parlamentari eletti gareggiando - uso questo termine non a caso